Signor Presidente, credo che la motivazione per il non passaggio agli articoli

necessario - meglio sarebbe dire era necessario vista la data di deposito del provvedimento - in quanto il sistema giustizia non era preparato a recepire gli effetti degli ultimi decreti delegati.

Devo dare atto al ministro Mastella di aver posto in essere oggi un estremo tentativo di mediazione. Il Ministro, che certamente è un politico,

fosse entrata in vigore. Ciò vale anche per qualcuno dei tre provvedimenti in discussione, soprattutto per quello che riguarda l'Ufficio del giudice.

a sanare situazioni di vera e propria anarchia esistenti in alcune procure. Abbiamo lavorato tutto il giorno, seriamente, credo tutti con spirito aperto, per trovare una soluzione, un accordo

dagli incontri e dai confronti di oggi è stata questa. Siamo tornati di nuovo al punto fondamentale. C'è una parte di questa maggioranza, che è formata soprattutto da ex magistrati - formalmente, in realtà, magistrati militanti ancora nello spirito e nella mente, anche se senatori - che non ha voluto arrivare ad un accordo. Ci deve essere uno scontro, perché quest'Aula deve essere teatro di uno scontro finale. La riforma Castelli deve essere cancellata in quanto vista come un *vulnus* al potere della magistratura. Bisogna ristabilire l'ordine delle cose per le quali da anni, anni e anni questo Parlamento in materia di giustizia non può legiferare se la magistratura non è d'accordo. Questo è il dato fondamentale con il quale noi oggi oggi dobbiamo ancora una volta misurarci. Credo che su questo gli stessi colleghi dell'attuale maggioranza dovrebbero meditare, anche se vedo che i giochi sono fatti. Consiglio a tutti la lettura di un libro interessante, «Il giudice sovrano», che ci dimostra come questa deriva dicastocratica, permettetemi questo termine, sia un fenomeno mondiale, che non riguarda soltanto il nostro Paese. Ma oggi la partita si gioca su questo tema e credo sia ancora aperta. Vedremo come

Non c'è riuscito. Era circondato, li ho contati, da ben otto magistrati o ex magistrati. Non so se anche lui, al pari del primo ministro Prodi, per il quale è stato chiesto un comitato di sostegno,

la proposta di non passare all'esame degli articoli non vuole essere una proposta meramente ostruzionistica, così come d'altra parte eravamo abituati nella scorsa legislatura, ma un'ultima possibilità di confronto e di dialogo. Signor Ministro, ho apprezzato molto la sua voglia di arrivare ad una mediazione, ad un confronto, però, me lo permetterà, è arrivato un po' in ritardo, perché se già da quando lei è venuto in Commissione giustizia avesse indicato delle linee di riferimento in relazione alla modifica dell'ordinamento giudiziario, se già sulla base di queste si fosse inaugurata in Commissione la possibilità di un confronto concreto e costruttivo anche sulla modifica, oggi non ci troveremmo in «zona Cesarini», strozzati strozzati dall'incombere dell'Aula. Soprattutto, avremmo potuto discutere con maggiore serenità e tranquillità. Avremmo potuto veramente lavorare assieme. Tutto ciò non è avvenuto. Solo in fase di replica lei ha indicato e ribadito una serie di linee di indirizzo. Ne ha discusso anche in sede di trattativa, ma tutto questo sembra frutto di una sollecitazione, di una rincorsa, di un voler dire: «noi qualcosa nel cassetto lo abbiamo».

riforma. Evidentemente tutto questo ha fatto perdere tempo e alla fine ci siamo ritrovati con una discussione nella quale sono emersi momenti particolarmente incisivi ed importanti. Credo, signor Ministro, che tutti concordino sulla necessità di evitare che l'azione disciplinare crei degli ingolfamenti e di rivederla in alcuni passaggi. Ci siamo però fermati su alcuni punti essenziali. Al di là, infatti, della circostanza che lei comunque ha affermato di condividere, ovvero della possibilità di ipotizzare la separazione delle funzioni

in proposito il collega Castelli probabilmente avrà anche pensato male, ma, come si suol dire, a pensare male forse ci si indovina, cerca a tutti i costi di condizionare la politica da fuori e di eterodirigerla. Ecco perché il ritorno in Commissione, il non passaggio agli articoli apre, in modo assoluto, lo scenario al confronto costruttivo su ogni punto, evidentemente con una prevalenza dell'indirizzo della maggioranza, perché questo è fin troppo evidente, il risultato elettorale è fuori discussione,

C'era un convitato di pietra, che forse era anche presente nell'aula in cui abbiamo trattato e discusso, che con i suoi *niet* tecnici o pseudo tali ha escluso, a fronte di una disponibilità che abbiamo percepito e che ci è stata manifestata da parte dell'elemento politico, la possibilità di arrivare non ad uno stravolgimento del vostro indirizzo, ma all'attuazione di un modo di intendere la giurisdizione, in particolare l'ufficio del pubblico ministero, in cui non è pensabile che vi possano essere difformità di indirizzo, in cui ci deve essere comunque un capo dell'ufficio che ovviamente va controllato nel suo operato, ma non dal Consiglio superiore della magistratura, non dall'assemblearismo, non dalle correnti,

in quel fascicolo, sottratto al pubblico ministero, l'ipotesi di un estremo d'azione disciplinare, ovvero per il procuratore come per il sostituto. tutto questo ci ha portato a irrigidimenti, al voler accogliere dei *totem*, perché tali sono per coloro che purtroppo hanno dimostrato di sapere condizionare e eterodirigere questa maggioranza. Alla fine, però, perde la politica; perde cioè la possibilità che la politica si confronti senza avere a cuore interessi dell'una o dell'altra categoria, ma avendo a cuore un sistema che funziona e in ordine al quale tutti si affannano a dire che oggi non funziona. Ne vogliamo parlare? Noi siamo pronti al dialogo, ma non certamente con termini giugulatori e con la possibilità che l'incombere della discussione in Aula limiti il dibattito e impedisca i ragionamenti, fuori e dentro il luogo della trattativa, che fanno parte dell'attività della politica.

il Gruppo UDC è particolarmente rammaricato per il fatto che, nonostante il tentativo, lungamente perseguito, di un'intesa politica su un fatto di regole istituzionali (come quello concernente l'ordinamento giudiziario), non sia stato possibile raggiungere

questo, perché abbiamo ripetutamente affermato, anche in quest'Aula, di essere favorevoli a cercare l'intesa sulle regole; ma, quando la nostra disponibilità è stata messa alla prova, purtroppo ci è stato detto che non era possibile. Prendiamo atto con molto rammarico di questa impossibilità. Ci auguriamo che in futuro la maggioranza si possa pentire seriamente di quanto ha fatto oggi.

poiché non credo che sia possibile oggettivamente prospettare ai cittadini italiani che una riforma quale quella dell'ordinamento giudiziario, che si attendeva da moltissimi anni, possa essere vanificata, *rectius* sospesa, con un atto di imperio dell'attuale maggioranza, su punti estremamente delicati e senza, peraltro, che vi siano delle norme transitorie che vadano a sanare le problematiche evidentissime. Sono infatti ormai entrate in vigore le parti della cosiddetta legge Castelli, che quindi verrebbe ad essere sospesa senza che a regime rimanga assolutamente nulla. nulla. La votazione sugli articoli è quindi assolutamente un fuor d'opera, quando pacificamente si poteva trovare un accordo tra maggioranza ed opposizione per addivenire ad un testo che fosse veramente più consono alle esigenze della magistratura e della cittadinanza. Vedete, bloccare ancora una volta la separazione delle funzioni, per cui chi è pubblico ministero il giorno dopo può andare a svolgere funzioni di giudicante, è una cosa straordinaria, che non è consentita in uno Stato di diritto e non è consentita dall'articolo 111 della Costituzione. Evitare, ancora una volta, che i procedimenti disciplinari abbiamo un'oggettiva tipizzazione è un qualche cosa che va al di là delle regole di diritto certe. Far sì che i concorsi vengano accantonati e si continui a procedere per anzianità è, anche questo, un fuor d'opera. Mi rendo conto delle pressioni straordinarie che il potere giudiziario sta esercitando sulla maggioranza; ma a me pare che questa sarebbe l'occasione, vista la disponibilità che è stata data da tutta l'opposizione, per poter addivenire a norme concordate, per fare una breve pausa di riflessione vera in pochi giorni, questi articoli. Mi pare straordinaria la tesi che non si sia in grado di apportare delle modifiche strutturali ad una legge che pacificamente è già in vigore. Vi sono stati anni e anni di discussione tra noi, nella passata legislatura, e mesi e mesi dalle ultime elezioni. Quindi, che ci si venga dire non è possibile, per l'attuale maggioranza, avanzare una proposta oggettiva sull'ordinamento giudiziario significa una povertà di contenuti e di programmi che lascia stupiti; salvo che, come diceva il senatore Castelli, non ci sia soltanto la volontà di porre nel nulla una riforma che è lungamente aspettata dal Paese. A me pare, quindi, che la sospensione della votazione degli articoli sia un atto dovuto, vista la disponibilità pacifica da parte di questa opposizione di arrivare ad un miglioramento di una legge che è già in vigore. del provvedimento in esame si appaleserà immediatamente; non so come potrà il Capo dello Stato firmarlo e far sì che vengano sospese delle norme già in vigore, senza che rivivano le norme precedentemente abrogate. Non ho, nella mia esperienza, mai visto una legge che preveda siffatto metodo e francamente non riesco a comprendere come si possa, anche con quei pannicelli caldi che sono gli emendamenti proposti dal Governo, addivenire ad un sistema che vada a regolamentare le norme pacificamente già abrogate.

nelle passate settimane il problema dell'utilità di una possibile trattativa fra le parti politiche e del valore di un eventuale risultato positivo di questa trattativa non era sfuggito al presidente del Senato del Senato Marini, il quale anzi aveva in qualche maniera operato in quella direzione, che oggi abitualmente si chiama di *moral suasion*, perché le parti si incontrassero e si potesse giungere ad un risultato di questo tipo. Il valore di questo risultato non deve sfuggire a nessuno: sarebbe stato un fatto assolutamente nuovo nuovo nel panorama politico e istituzionale del nostro Paese, un messaggio assolutamente innovativo, assolutamente originale nei confronti dei cittadini, abituati ormai da decenni a vedere le parti politiche del Paese contrapposte fra di loro sul tema della giustizia, se - pur ferme le posizioni di ciascuno in termini di principio

offrire alla comunità dei cittadini. Non siamo riusciti a pervenire ad un risultato, malgrado le componenti della Casa delle Libertà abbiano accettato di rinunciare alla critica di fondo, alla critica di scenario che avevano avanzato quando il Ministro della giustizia aveva proposto il disegno di legge di cui stiamo discutendo. Avevamo allora detto, questa primavera, all'inizio dei nostri lavori della XV legislatura, che se il Ministro, se il Governo, se l'attuale maggioranza condiviso in tutto o in parte la riforma che passa sotto il nome di riforma Castelli, avrebbero potuto proporre un disegno di legge che la modificasse in tutto o in parte, paradossalmente che la sopprimesse. Il ministro Mastella più volte ci ha ripetuto che non era questo il suo intendimento, né quello dell'azzeramento della riforma, né quello dell'annullamento o della controriforma di qualche misura. ministro Mastella ci ha più volte ripetuto che egli intendeva, attraverso lo strumento della sospensione, eliminare qualche criticità

l'ufficio del pubblico ministero e la sua riorganizzazione secondo un modello assolutamente innovativo, il processo disciplinare, invocato a parole dai magistrati ma che domani, quando questo disegno di legge - se la maggioranza sarà presente - sarà votato, sarà ancora una volta azzerato e infine il sistema dell'accesso in magistratura e dei concorsi. Nelle riunioni di questa mattina e di questo pomeriggio - credo che se ne debba dare pubblico atto - ci siamo confrontati allo scopo principale di far emergere queste criticità.

(decreto-legislativo che è in vigore da ormai 7 mesi e che, possiamo ragionevolmente ritenerlo, resterà in vigore per almeno un anno, considerando i tempi che occorreranno dopo che il disegno di legge passerà dall'esame

dell'accesso alla magistratura e dei concorsi. Abbiamo, in definitiva, proposto che, laddove non siano state riscontrate criticità, non occorre sospendere nulla. Sarebbe, anzi, un'indicazione assolutamente distorsiva quella di

Abbiamo, viceversa, convenuto che, laddove esistano delle criticità, saremmo stati disponibili a intervenire con correzioni concordate in tempo reale, destinate a migliorare il risultato concreto che, in definiva, è proposto agli operatori e ai cittadini, ovvero di procedere alla sospensione. Su questo punto, signor Presidente, le nostre discussioni si sono arrestate sulle seguenti parole: per noi l'aggettivo «esclusivo» è un *totem*. Lei capisce bene, signor Presidente, che di fronte ai *totem*, non si può dialogare:

Va rispettato, va infranto quando ve ne è la possibilità e la condizione (in questo caso la condizione è politica), ma non può essere oggetto di dialogo. Oggi noi abbiamo responsabilmente offerto e il presidente Marini ha responsabilmente offerto alla sua maggioranza (ma egli ha mostrato di essere in questa circostanza senz'altro il Presidente di tutti senatori) di tutti senatori) la possibilità di smarcarsi rispetto a quello che è stato chiamato il «convitato di pietra», piuttosto che quello che è stato chiamato il

credo che, attraverso la ridiscussione del disegno di legge in Commissione e il non passaggio agli articoli, si possa mantenere aperto questo spazio opportuno che il Presidente del Senato ha voluto offrire a tutti noi.

in dichiarazione di voto per chiedere all'Aula il voto favorevole alla proposta di non passaggio agli articoli illustrata dal presidente Castelli.

in questo modo l'efficacia dei decreti legislativi, si crea una grave confusione nell'ordinamento giudiziario e

Dopo molte ore di discussione, il senatore Castelli - forse stanco - si è accorto del comitato di controllo di magistrati intorno al ministro Mastella,

esercitasse l'azione penale delegandola ai suoi sostituti e, nel caso di rottura degli accordi o di contrasto, fosse previsto il ricorso al Consiglio superiore della magistratura. La Casa delle Libertà, invece, voleva che questo ricorso andasse al procuratore generale, causando così uno stravolgimento dell'ufficio, all'interno del quale, con l'attribuzione di poteri veramente impropri al procuratore generale, ci sarebbero stati due capi

di un corretto uso di questo potere, né stravolgendo l'ordinamento giudiziario in uno dei suoi punti fondamentali. Quindi, io sono d'accordo

Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo fatto tutto il possibile per avviare subito un confronto serio sulle norme in materia di ordinamento giudiziario, essendo convinti che l'ordine giudiziario e il sistema giustizia abbiano bisogno di nuove norme, quanto più possibili condivise, in materia di ordinamento giudiziario. il nostro atteggiamento in questi giorni è stato di chi tende la mano per trovare già adesso una possibile intesa sul disegno di legge in discussione, che sospende le norme delegate, sulle proposte e sui progetti da tradurre quanto prima possibile in norme di legge. Abbiamo voluto l'incontro di questa mattina e abbiamo voluto la discussione di merito svolta in queste ore, avanzando la proposta di salvare alcune delle norme dei decreti Castelli. L'intendimento politico era quello di dare un segnale all'opposizione: facciamo scemare il contrasto, cerchiamo un punto di incontro e poi lavoriamo assieme, anche abbreviando i tempi della sospensione, per arrivare prima alla definizione di norme sull'ordinamento giudiziario che possano raccogliere un consenso più ampio rispetto ai limiti della maggioranza di Governo. Governo. Sul decreto che si riferisce ai concorsi, su quel meccanismo complesso che ha suscitato riserve e che anche voi ritenete

pur convenendo sostanzialmente sulle linee di una modificazione delle norme Castelli, di fermarci e di lavorare con maggiore capacità di riflessione e con tempi non strettissimi.

È evidente che quando si vuole stabilire, come voi avete proposto fino all'ultimo, creando da parte nostra delle difficoltà, che sia il procuratore generale a decidere sulla revoca del procedimento e sull'eventuale contrasto insorto tra sostituto e procuratore della Repubblica, allora si introduce

nell'ambito di questo dibattito di una posizione di critica più radicale rispetto alle nostre proposte, che non è soltanto per ragioni funzionali che abbiamo voluto e vogliamo la sospensione dei decreti delegati. Non è solo perché il Consiglio si è appena rinnovato, non è soltanto per superare difficoltà organizzative che è stato presentato il disegno di legge di sospensione; o meglio, vi sono ragioni di funzionalità, ma vi sono anche ragioni di funzionalità derivanti da norme che a nostro avviso sono sbagliate. Per quello che riguarda le norme in materia di responsabilità disciplinare, se s'introduce l'obbligatorietà dell'azione disciplinare senza stabilire un filtro, un potere di archiviazione per l'irrilevanza dei fatti, si porta il sistema al collasso; nei procedimenti disciplinari un intervento di un delegato del Ministro accanto alla procura generale è, a nostro giudizio, norma non accettabile. Allora, noi non condividiamo questi aspetti delle norme sull'ordinamento giudiziario; abbiamo voluto la sospensione per poter costruire insieme, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nuove norme più soddisfacenti che siano anche sottratte allo scontro che ha accompagnato la politica della giustizia nella scorsa legislatura. Si dice che occorre legiferare indipendentemente dalle spinte particolari; ho sentito parlare qui di convitati, di un comitato che circonda il Ministro e che sarebbe portatore di interessi particolari. Sono letteralmente stupefatto, perché abbiamo visto giocare nella preparazione e nell'approvazione di leggi in tema di giustizia interessi particolari; lo abbiamo visto nella scorsa legislatura, nelle leggi che non abbiamo condiviso, che abbiamo criticato e che a tutti i costi la maggioranza ha voluto imporre al Parlamento. Allora, non trascinateci per i capelli verso la riapertura di una polemica che non conviene a nessuno e che non aiuta il nostro lavoro. Non ci sono interessi particolari che dettino le nostre scelte qui: c'è una concezione dell'ordinamento giudiziario che evidentemente non corrisponde alle idee guida dei decreti delegati, almeno per certi aspetti. Quindi, noi diciamo di ridiscutere insieme; è possibile - per quello che ho sentito anche nella riunione di oggi - trovare punti d'intesa comune; abbassiamo dunque il tono delle polemiche e cerchiamoli. Per far questo, però, la maggioranza ritiene che la sospensione dei decreti - avremmo voluto una sospensione parziale, non siamo riusciti a trovare questa intesa - ci consenta un lavoro serio e un confronto nel merito. Ho ascoltato con attenzione, e lo ringrazio, il collega D'Onofrio, il cui intervento è stato tra i più pacati nella discussione di pochi minuti fa; penso che sia possibile la convergenza, sulla base di quel che ho ascoltato nel suo intervento, che dobbiamo cominciare a costruirla dobbiamo cominciare a costruirla subito, che già un pezzo - piccolo purtroppo - di cammino lo abbiamo fatto nella giornata di oggi. Per questo, noi chiediamo ai colleghi, a tutti i colleghi - l'opposizione naturalmente si regolerà

e che rifiuta la pausa, la riflessione che invece noi riteniamo indispensabile al confronto. Per questo voteremo contro il non passaggio all'esame degli articoli e dalle prossime ore siamo pronti al confronto in Commissione giustizia, fuori da essa, nel dibattito nel dibattito che deve aprirsi per arrivare al più presto possibile - ben prima del mese di luglio - a definire norme nuove su quelle materie dell'ordinamento giudiziario rispetto alle quali abbiamo sospeso l'efficacia dei decreti delegati.

individuazione delle ragioni a base degli emendamenti, poiché si tratta di tre decreti delegati tutti concentrati sull'articolo 1, cui sono riferiti la maggior parte degli emendamenti presentati, trattandosi di materie assolutamente differenti,

ricompreso nell'articolo 1, piuttosto che fare un discorso assolutamente generale e omnicomprensivo.

esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che, secondo i chiarimenti forniti dal Governo, dalla sospensione delle norme già in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, non derivano conseguenze negative sul bilancio dello Stato, non avendo le norme stesse, ad oggi, prodotto effetti di carattere finanziario. Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.12, 1.24, 1.23, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.334, 1.99, 1.335, 1.100, 1.336, 1.101, 1.337, 1.102, 1.103, 1.104, 1.338, 1.105, 1.339,

1.347, 1.137, 1.348, 1.349 e 1.350, sulle quali il parere è contrario, nonché delle proposte 4.5, 4.301, 4.6, 4.7 e 4.8, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione». Onorevoli colleghi, a norma dell'articolo 97 del Regolamento, sono improponibili gli emendamenti estranei all'oggetto del disegno di legge che, in questo caso, concerne la sospensione dell'efficacia delle disposizioni recate dai decreti legislativi nn. 106, 109 e 160, nonché di alcune altre norme ad essi collegate. La Presidenza ritiene pertanto ammissibili unicamente gli emendamenti diretti a modificare il termine di sospensione ovvero a limitarlo a uno o più decreti legislativi, ovvero a modularlo differentemente per i singoli decreti. Ritiene altresì ammissibili gli emendamenti diretti a limitare gli effetti della sospensione a singole parti dei decreti legislativi, a condizione che essi non incidano sull'impianto normativo complessivo del decreto legislativo in questione, in modo da determinarne o una surrettizia modifica nel merito ovvero una sostanziale inapplicabilità. Risultano invece improponibili gli emendamenti 1.12, 1.24, 1.23, 1.35, 1.317, 1.37, 1.318, 1.26, 1.38, in quanto sospendono l'efficacia dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, consentendo però l'immediata applicazione o la modificazione del termine di sospensione di altre disposizioni del decreto esplicitamente correlate all'articolo 1 stesso. Sono altresì improponibili gli emendamenti da 1.46 a 1.59, in quanto ognuno di essi sospende l'efficacia, con effetti del tutto incomprensibili, di singole fattispecie incolpatrici tra quelle previste dalla tipizzazione degli illeciti disciplinari recata dal decreto legislativo n. n. 109 del 2006. Sono improponibili gli emendamenti 1.326, 1.95, 1.96, 1.97, 1.102, 1.103, 1.118, 1.409, 1.410, 1.411, 1.412, 1.414, 1.416, 1.419, 1.420, 1.426, 1.431, 1.432, in quanto determinano l'applicazione immediata di disposizioni recate dai singoli decreti legislativi che fanno riferimento esplicito ad altre disposizioni dei medesimi decreti la cui efficacia viene invece sospesa. Sono, infine, improponibili gli emendamenti 3.301, 4.0.300, 4.0.301, 4.0.302, 4.0.303, in quanto apportano modifiche di merito ai decreti legislativi in questione, alla legge delega o ad altri decreti legislativi in materia di ordinamento giudiziario.

Senatore Caruso,

Se non mi è sfuggito nella sua rapida lettura il passaggio relativo a questo emendamento, ho compreso che esso è ritenuto dal Presidente del Senato pertinente, compatibile e non esorbitante dall'impianto del disegno di legge

voglio richiamare l'attenzione su questo singolare balletto della proponibilità e della improponibilità degli emendamenti. Conosciamo tutti bene la norma di Regolamento da lei, signor Presidente, richiamata, talmente bene da sapere anche perfettamente in quale maniera la stessa sia stata tradizionalmente, storicamente applicata dall'Aula del Senato e, di conseguenza, dalle Commissioni del Senato. Sappiamo perfettamente come l'applicazione della stessa abbia avuto particolare rigore con riferimento alle leggi di conversione di decreti-legge e attenuato, attenuatissimo, inesistente rigore con riferimento ai disegni di legge ordinari, quale è quello al nostro esame. Quando tale provvedimento si è affacciato ai lavori della Commissione si è posta immediatamente la questione della improponibilità o proponibilità di taluni emendamenti. Il presidente Salvi ritenne, sospendendo per questa ragione i lavori della Commissione, di sottoporre la questione al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato comunicò un'interpretazione non restrittiva, ma restrittivissima della norma di Regolamento di cui oggi si discute, per la prima volta applicata

all'ultimo dei controversi decreti‑legge di cui si è occupata quest'Aula e mi riferisco al decreto-legge Bersani. Tutti noi sappiamo benissimo che il decreto-legge Bersani è entrato in quest'Aula in una certa maniera e sappiamo benissimo che ne è uscito arricchito - ad uso degli

disciplina il sistema di proponibilità o improponibilità degli emendamenti. In questa occasione, per la prima volta il Presidente del Senato torna alla più stretta, strettissima ortodossia e, con riferimento all'emendamento 3.600 (testo 2) del Governo, contraddice, signor Presidente, se stesso. Questo emendamento è assolutamente distante, assolutamente estraneo alla volontà legislativa contenuta nel disegno di legge e, quindi, la invito, signor Presidente, a riconsiderare la sua decisione e a dichiararlo improponibile.

ma la sospensione di una norma relativa alla legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura e in particolare il rientro in ruolo dei consiglieri superiori uscenti. uscenti. Signor Presidente, quando si ritiene, come è scritto nel disegno di legge, di dover modificare quella norma, vale a dire l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica abrogando implicitamente, sia pure temporaneamente, una disposizione del 2002 per fare rivivere una precedente disposizione del 1958, e si assume che questa disposizione dev'essere in vita, previa sospensione delle altre, fino al 31 luglio del 2007 (con buona pace del senatore Brutti che poc'anzi faceva riferimento a leggi *ad personam*), sostanzialmente si crea una legge *ad personas* che riguarda i sedici componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. Signor Presidente, vorrei capire la ragione per la quale viene dichiarato improponibile un emendamento che riguarda specificatamente la disciplina del rientro in ruolo dei consiglieri superiori uscenti, quando nel disegno di legge si consente di modificare quella disciplina attraverso la sospensione di una norma del 2002 che, essendo protratta per un anno, consente ai sedici consiglieri superiori uscenti di giovarsi della precedente normativa. Davvero non riesco a comprendere le ragioni di questa improponibilità.

capisco che è prevista anche la riammissione in ruolo in caso di soprannumero. Vorrei ricordare che questo tema è stato ampiamente dibattuto in sede di approvazione della riforma e che la Presidenza della Repubblica ha sempre dichiarato che il soprannumero era inammissibile per motivi costituzionali, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

caso di risposta negativa, come presumo, ci dovrà essere una votazione elettronica, perché l'Aula deve votare su un emendamento che patentemente non ha copertura finanziaria.

la parte assolutamente pregnante del provvedimento è l'articolo 1. Forse sarebbe stato meglio suddividerlo per argomenti, visto che comprende

i parenti non possano operare nello stesso ufficio, qualunque esso sia. Questa norma vale per tutti gli italiani, vale per tutti gli uffici, ma non vale per un'unica categoria: i magistrati.

Signor Presidente, non sono riuscito, e l'ho già confessato, a prendere debitamente nota di tutti gli emendamenti dichiarati improponibili e segnatamente dei miei, né ho la lista, che non è stata posta a disposizione dei senatori o quantomeno non è pervenuta a me. Questo mi impedisce di illustrare puntualmente emendamento per

sul fatto che, per esempio... Come dicevo, gli emendamenti da me proposti intervengono in una prima area, quella della proposta di non procedere alla sospensione di alcuni dei decreti delegati ormai in vigore, vigore, naturalmente come ipotesi subordinata rispetto a quella di non sospenderne alcuno e quindi, in definitiva, di rinunciare alla parte centrale del proposito normativo. Con riferimento a ciascuno dei tre decreti delegati oggi in vigore, devo ricordare che quello che riguarda il pubblico ministero, ad esempio, è uno strumento normativo - di cui è chiesta la sospensione - composto solamente da otto articoli.

dei primi. Signor Presidente, sospendere questo decreto legislativo, affermando che non si vuole dare luogo all'azzeramento della riforma, ma che si vuole semplicemente procedere alla futura e ragionata modifica della riforma riforma stessa, proposta dal Governo di centro-destra nella XIV legislatura, è - non me ne vogliano i colleghi e non me ne voglia lei, signor Presidente - una marcata, una dichiarata, una non revocabile in dubbio grande ipocrisia.

dei decreti legislativi e non di tutti e tre, come il Ministro ha proposto, riguarda, ad esempio, il decreto legislativo n. 109 del 2006, in materia di

condivisibilità. Non posso pensare che il ministro Mastella o la maggioranza di centro-sinistra vogliano non condividere il principio enunciato già solo nell'articolo 1 della prima sezione del Capo I del decreto legislativo, che parla dei doveri dei magistrati. Posso immaginare che il ministro Mastella, che parte della maggioranza, che l'intera maggioranza attuale non condivida il catalogo

mi sembrano assolutamente non revocabili in dubbio. Apro una breve parentesi, signor Presidente. Nella XIV legislatura ho avuto l'onore di presiedere la Commissione giustizia; so bene come sono nate queste norme, ne conosco non solo i momenti immediatamente formativi, ma anche i momenti mediatamente formativi. Ritengo di poter essere creduto, come memoria storica su questo punto, se dico che nel catalogo dei disvalori

Pertanto non posso credere che tutto questo apparato debba essere necessariamente sospeso. Né posso credere che si vogliano revocare in dubbio le scansioni della sanzioni, come sono contenute nella seconda sezione del decreto decreto legislativo, e la relativa didascalica esplicazione. Allora mi domando: che necessità vi è di sospendere uno strumento complesso, che è un valore aggiunto consegnato ai cittadini? Questi oggi sanno che anche chi li giudica non è immune da giudizio; anche chi li giudica, anche chi ha lo smisurato potere di privarli della libertà può, a sua volta, essere giudicato, non peraltro al di fuori della sua *enclave*. Dobbiamo infatti ricordare che giudice dei giudici restano i giudici, attraverso il Consiglio superiore della magistratura. Perché eliminare questo valore aggiunto di democrazia e trasparenza che è stato consegnato ai cittadini? Perché procedere ancora una volta ad una ipocrita sospensione? Sono perfettamente consapevole - l'ho detto senza infingimenti in ogni sede, parlamentare e non parlamentare

Perché il ministro Mastella non rinuncia a sospendere questo decreto legislativo lasciandolo in vigore e affidando, ad esempio, ad un decreto-legge, che certamente avrebbe le caratteristiche costituzionali dell'urgenza e della necessità, quegli interventi modificativi e perfezionativi

una qualsiasi senatore, ma da un organo costituzionale, qual è il Consiglio superiore della magistratura?

635. Credo di aver rassegnato all'Assemblea le ragioni per le quali ho presentato un complesso di emendamenti, alcuni più fortunati, altri meno, a seconda delle novità introdotte dal presidente Marini nella determinazione dell'improponibilità, che mirano a suggerire al ministro Mastella o di non intervenire attraverso lo strumento della sospensione, fermo il suo intangibile diritto di intervenire attraverso lo strumento della modifica ed anche dell'abrogazione, ovvero a proporre al ministro Mastella, al Governo ed alla maggioranza di centro-sinistra di intervenire nella maniera da loro scelta, ma con un provvedimento a geometria variabile, che lasci sane le parti che non hanno alcuna ragione di essere immediatamente modificate attraverso una misura di sospensione. Si sospende quello che procura danno, ma ancora non abbiamo sentito dire dal Ministro ciò che procura danno, con riferimento almeno ad una parte significativa dei tre decreti legislativi.

CASSON *(Ulivo)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la sospensione dell'articolo 1 tocca il cuore della discussione che dobbiamo affrontare. Il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, fa riferimento sostanzialmente al problema della gerarchizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, un'impostazione della procura della Repubblica che ci vede nettamente contrari. 20 febbraio 2006, n. 109, riguarda l'azione disciplinare, così com'è stata impostata dalla riforma Castelli, con un'azione disciplinare obbligatoria e la tipizzazione degli illeciti disciplinari.

e alla separazione delle funzioni requirenti e giudicanti. Intendiamo arrivare alla sospensione di tale riforma per una questione fondamentale. Così come ha avuto modo di riferire il Ministro

ciò che soprattutto non accettiamo è l'impostazione della figura del procuratore della Repubblica come titolare esclusivo dell'azione penale:

l'esclusività dell'azione penale. La questione riguarda le assegnazioni dei fascicoli, il potere assoluto di revoca e persino la possibilità di decidere

per poter pervenire a un testo condiviso. Abbiamo verificato che tale volontà in realtà non c'era, ma permaneva invece il tentativo di reinserire la gerarchizzazione degli uffici del pubblico ministero:

certune fattispecie che devono essere affrontate in maniera più dettagliata. In questo momento è anche tecnicamente sbagliato procedere ad una sorta di "riforma arcobaleno", intervenendo su questo decreto legislativo

soprattutto per il periodo transitorio, va comunque prospettata una sorta di filtro, che va approfondito nella sede adeguata. Gli effetti del decreto legislativo n. sono gravi, perché, come ha avuto modo di dire in altra sede l'attuale Vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, questa impostazione rischia di portare a un blocco dell'attività della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Ciò significa, al contempo, fare arrivare verso la prescrizione tutti i procedimenti pendenti e quelli che si possono innestare, vista la prescrizione estremamente limitata inserita all'interno di questo decreto della riforma Castelli. Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 160, gli aspetti che ci preoccupano sono ancora maggiori. Si tratta, forse, del cuore della riforma,

che si prospetta definitiva, si crea una situazione piuttosto grave per la progressione e la possibilità per il magistrato di operare all'interno della magistratura in una funzione o nell'altra. Proprio per evitare

siamo contrari agli emendamenti perché, ovviamente, porterebbero ad una riaffermazione della validità della

decreto legislativo, forse il più importante, tanto che proprio su di esso oggi si è determinata una rottura nella faticosa trattativa per cercare di arrivare ad un voto condiviso sui tre decreti legislativi. La riforma Castelli dell'ufficio del pubblico ministero ha ignorato l'articolo 107 della Costituzione, il quale al terzo e quarto comma afferma che: «I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario». Si prefigura in

Non c'è dubbio che così come il giudice è sottoposto soltanto alla legge, nello stesso modo anche il pubblico ministero è sottoposto soltanto legge e non può essere sottoposto alla gerarchia. Invece, con la riforma Castelli si ipotizzava un ufficio gerarchico, al punto che il *dominus* dell'azione penale, dalla sua genesi alla sua fine, era solo e soltanto il capo dell'ufficio. Noi contrastiamo questa idea perché ci riporta indietro indietro ad anni molto bui di questa Repubblica. Forse, abbiamo dimenticato gli anni della procura di Roma e del cosiddetto porto delle nebbie, gli anni in cui il CSM aveva una legge elettorale maggioritaria, ragion per cui un gruppo di magistrati minoritari riusciva a conquistare tutti e 20 i seggi del Consiglio superiore, così anche la scelta dei procuratori della Repubblica e dei capi degli uffici. All'interno di quel Consiglio superiore

come si diceva una volta, che i giudici erano servi del potere. Non è vero, in quanto i giudici condividevano in pieno l'ideologia del potere; facevano le stesse scelte ideologiche, le stesse opzioni culturali, provenivano dagli stessi ambienti. Essi erano espressione di quella stessa classe che poi esprimeva il potere di Governo. Ecco perché siamo contrari Non possiamo tornare indietro, Non possiamo tornare indietro, alla procura della Repubblica di Roma dove tutto veniva insabbiato. Dobbiamo guardare avanti e sempre e soltanto alla luce della Costituzione repubblicana.

di riferire al presidente Marini. Abbiamo fatto un accordo, in sede di Conferenza dei Capigruppo, un accordo che intendiamo rispettare.

vorrei se ne tenesse conto perché, lo dico senza malizia, ho l'impressione che da parte della maggioranza

che comunque la sua eccezione sia fondata perché - per chi non è avvezzo alle regole del Senato - avendo fissato l'orario entro cui concludere l'esame degli articoli e la votazione finale e non avendo proceduto al contingentamento dei tempi - quindi alla distribuzione per i singoli Gruppi - paradossalmente qualcuno potrebbe prendere la parola da

- anzitutto per l'autorevolezza della sua persona - una precisazione. Non stiamo facendo ostruzionismo; se l'opposizione avesse avuto la volontà di votare, sarebbe stato sufficiente non iscrivere tante persone a parlare. Siccome, signor Presidente, abbiamo scelto nella giornata di oggi la strada - per iniziativa del Governo, ma ovviamente anche per volontà della maggioranza di attivare il dialogo, per quanto possibile, abbiamo ritenuto potesse essere sconveniente dare l'idea di non avviare - almeno sui primi emendamenti - un minimo di interlocuzione. Ora, essere accusati, perché volevamo interloquire e avviare un minimo di dialogo, di voler fare, noi, ostruzionismo al voto, mi pare francamente improprio. Assicuro, tuttavia, il presidente Matteoli che non parleremo più. Tuttavia, per quelli che ci ascoltano e per l'opposizione, a questo punto comprenderà che il nostro atteggiamento in qualche modo deriva anche da questi rimproveri cortesi che ci vengono mossi, per cui mi auguro che non parli non solo la maggioranza, ma nemmeno l'opposizione. In tal modo, signor Presidente, voteremo rapidamente, come lei

di non far sì che tutti gli emendamenti che non fossero stati votati alle ore 15 di domani debbano decadere e cercare di procedere nei nostri lavori con celerità ed equilibrio negli interventi, non privando l'Assemblea della possibilità di votare gli emendamenti

in relazione alla sua ultima affermazione, vorrei ricordare come nella Conferenza dei Capigruppo non si sia stabilito il principio, da lei evocato poc'anzi, della decadenza automatica degli emendamenti. È stato fissato un accordo reciproco reciproco che prevedeva un'intesa: il voto finale per la giornata di martedì pomeriggio e la chiusura del voto degli emendamenti nella giornata di giovedì. Non è stato fissato un orario; non vi è quindi una decadenza automatica. Era prevista una seduta fiume per la giornata di giovedì. Questo era l'accordo stilato nella Conferenza dei Capigruppo e non una decadenza automatica. Riallacciandomi - seppur brevemente - all'intervento del collega Matteoli, vorrei ricordare ai colleghi della maggioranza come

profondamente nel merito delle proposte. Nessuno può pensare né affermare, né nella maggioranza né nell'opposizione, che stamattina si sia dato luogo ad un confronto sterile e riduttivo. Non abbiamo trovato un'intesa, ma finalmente si è parlato di merito della proposta. Detto questo, invito la Presidenza di turno a rivolgere al presidente Marini una richiesta di convocazione della Conferenza dei Capigruppo perché in quella sede, possibilmente, in assenza di un accordo unanime di Assemblea che forse in questo momento non c'è, si possa rivisitare la possibilità di far scivolare di alcune ore il voto finale alla mattina di mercoledì proprio per ridare all'Assemblea la serenità di un dibattito compiuto che - confermiamo - non vogliamo caratterizzare con atteggiamenti ostruzionistici di alcun genere, ma soltanto con un confronto serio sui contenuti.

la finalità suprema di questo disegno di legge, afferma che l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legislativi nn. 106, 109 e 160

articolo portante di tutta la strategia che soggiace al disegno di legge sospensivo. Ebbene, avendo discusso, sia al momento della

dei decreti legislativi di cui trattiamo, credo che affermare con forza, da parte nostra, la necessità della soppressione di questo articolo, con cui chiudere la parte più

di diritti di libertà fondamentali per la cui tutela è sempre fatto riferimento all'autorità giudiziaria e a norme di garanzia. Ora, i decreti dei quali si chiede la sospensione riguardano proprio l'organizzazione giudiziaria e in particolare l'individuazione dei soggetti che esercitano la giurisdizione.

il principio secondo il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Il giudice naturale è quello indicato nelle norme dell'ordinamento giudiziario e nelle norme processuali. Aggiungo, inoltre, che vi sono norme del decreto legislativo relativo agli illeciti disciplinari dei magistrati che incidono sulla libertà degli stessi - libertà di associazione, libertà di parola e così via - e quindi vengono a impingere in maniera precisa con gli articoli

segreto, nessuno ebbe nulla da ridire e il presidente Fisichella, una garanzia per il suo stesso percorso politico *bipartisan*, concesse il voto segreto senza difficoltà.

vorrei rappresentarle che in uno dei decreti di cui si chiede la sospensione è previsto espressamente che la richiesta di misura cautelare, quindi un provvedimento strettamente incidente sulla libertà personale dei cittadini, debba essere preceduta dal visto del procuratore della Repubblica. Ciò equivale a dire, signor Presidente, che se per ipotesi si

Signor Presidente, a sostegno di quanto dicevano i colleghi, posso anche dire che nel decreto delegato relativo alla tipicizzazione degli illeciti disciplinari, vi è una serie di norme che fanno divieto di iscrizione ai partiti, e questo certamente incide sulla problematica di uno dei diritti fondamentali stesse norme contengono anche il divieto di partecipazione a manifestazioni organizzate da partiti o da altri, e anche questo incide su una delle libertà fondamentali garantite e tutelate dalla Costituzione. Questa rapida esemplificazione dà conto di una serie notevole di norme contenute nei decreti delegati che comunque incidono su tali diritti fondamentali. L'elenco sarebbe lungo e se si avesse tempo anche solo di esaminarlo tutto penso che ci troveremmo di fronte ad alcune decine di ipotesi tutte rientranti nella norma.

senatore Castelli, e a tutti coloro che hanno posto la questione. L'articolo che regolamenta il voto segreto fa riferimento alla complessità e al peso, all'interno di tale complessità, delle varie materie

grande simpatia per lei, ma l'argomento che ha scelto è assolutamente controproducente. Infatti, se nel complesso delle cose ci sono più fatti che attengono ad un rapporto che può essere squilibrato a seconda non solo dell'interpretazione ma anche dell'applicazione di una norma che riguarda una condizione soggettiva e un rapporto tra questa condizione soggettiva e la collettività, lei ha detto una cosa che aggiunge il plurale al singolare richiesto dal collega Brutti. Mi sembra che la sua fresca intelligenza le consenta di capire qual è la contraddizione.

relativa ad una norma che incideva su un diritto costituzionalmente garantito o meglio sul suo esercizio. una norma che, in conformità con la Costituzione, tendeva a regolare l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito da parte dei magistrati. La questione rispetto alla quale ciascun senatore doveva pronunciarsi riguardava la determinazione dell'ampiezza dell'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, quindi la limitazione di determinate facoltà rientranti nel diritto del magistrato come cittadino. Si può parlare qui di esistenza o inesistenza di facoltà rientranti in un diritto costituzionalmente garantito.

a dire della sospensione temporanea dell'efficacia di norme e quindi non si incide sull'attribuzione e sul riconoscimento di diritti. Il nostro voto incide sull'efficacia, subito o tra qualche mese, di un complesso di norme, neanche di una norma specifica specifica relativa all'iscrizione dei magistrati ai partiti o alla partecipazione a movimenti e associazioni. Per questa ragione il principio della tutela costituzionale non entra in gioco. Noi infatti ci limitiamo a decidere che queste norme

desidero svolgere un'osservazione sulla sua decisione ed una sull'intervento del senatore Brutti. Sulla sua decisione, che spero non sia definitiva,

è poi un'argomentazione ulteriore. Ammesso e non concesso che si volesse adottare il criterio di una percentuale rispetto all'estensione della norma sulla quale viene richiesta la segretezza, vi è un indubbio peso specifico che ha un'incidenza diretta sulla libertà dei cittadini. L'ordinamento giudiziario riformato riformato - piaccia o meno, ma non stiamo discutendo di questo - accentua la gerarchizzazione degli uffici di procura conferendo una responsabilità maggiore nella direzione dell'ufficio al procuratore della Repubblica. A me non sembra di secondo piano secondo piano e soprattutto priva di incidenza diretta sulla libertà di ciascuno di noi, la circostanza che la firma del procuratore della Repubblica, vale a dire la sua condivisione di una richiesta che a che fare con la libertà personale non sia qualcosa che essa stessa ha diretta incidenza sulla libertà personale. Per questo il voto riguarda i diritti di libertà dei cittadini, al di là che esso incida, anche soltanto per l'1 per cento, sull'intero complesso delle disposizioni di cui viene chiesta la sospensione. L'intervento del senatore Brutti necessita di appena qualche secondo di replica. Dice il senatore Brutti, se ho ben inteso la sua argomentazione, qui non stiamo disponendo un mutamento definitivo della disciplina, ma semplicemente una sospensione della sua efficacia. Sì, ma i diritti di libertà comunque conoscono un'incidenza nella parentesi interessata dalla sospensione. Quindi mi pare che coloro che ne subiranno una lesione in quel periodo comunque abbiano voce in capitolo per chiedere che il Parlamento possa esprimersi nella sua piena libertà.

essendoci il precedente rispetto all'emendamento presentato a suo tempo dal senatore Brutti, visto che il Regolamento mi dà la potestà di sentire la Giunta per il Regolamento, intendo farmi dare un aiuto in questo senso, proprio per verificare, e chiedo anche l'ausilio del presidente Salvi,

il nostro Regolamento prevede sia formulato in forma scritta proprio per dare la possibilità agli uffici e alla Presidenza di valutare la ricevibilità della richiesta senza dover sospendere dell'Aula e convocare la Giunta per il Regolamento. Se successivamente vi saranno altre richieste, vi pregherei che fossero già consegnate alla Presidenza. In merito ai quesiti, io credo che, rispetto all'emendamento interamente soppressivo, debba essere fatto valere il comma 7 dell'articolo 113 del Regolamento laddove dice: «Sulla prevalenza decide il Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento»,

non prevalente la parte da sottoporre a voto segreto, voteremo gli emendamenti interamente soppressivi in forma palese o con lo scrutinio elettronico, se verrà richiesto. Laddove vi saranno invece emendamenti che puntualmente andranno ad interessare le lettere degli articoli 2 e 3, dove si fa un evidente riferimento ad una limitazione delle libertà costituzionalmente tutelate, se vi sarà la richiesta, intendo autorizzare il voto segreto.

lei stesso ha avuto delle perplessità prima di prendere la decisione di non accedere alla richiesta del collega Pastore.

maggioranza ci poteva essere la richiesta di accedere favorevolmente a ciò che il collega Pastore aveva chiesto. Egli, infatti, non aveva chiesto di non votare, di cancellare un provvedimento, ma soltanto di esprimersi attraverso il voto segreto.

Resta il punto della sua decisione, che rispettiamo, ma resta anche questo aspetto politico che volevo sottolineare.

di allora era composta da decine di deputati - sulla questione pregiudiziale da me presentata, che riguardava appunto quella parte della legge delega concernente la riorganizzazione delle procure con un particolare riguardo a un principio costituzionale che è quello dell'obbligatorietà dell'azione penale e dei suoi riflessi sui diritti di libertà, mi fu negato il voto segreto e il provvedimento venne votato a voto palese.

Senatore Carrara chi c'è di fianco a lei? Calma, è aperta la votazione. Senatore Cantoni, dietro di lei c'è una luce alla quale non

le tessere da una parte e dall'altra che non abbiano il corrispondente, per cui se vi sedete controllo, diversamente... Uno alla volta, una l'abbiamo tolta, adesso procediamo con le altre. Colleghi, io non ricevo nessuna segnalazione se non dal Capogruppo e gli altri stiano seduti. Tornate a posto, colleghi. Almeno i Capigruppo mi diano una mano nello stare al posto ed eventualmente segnalare eventuali irregolarità

Presidente, lei ha perfettamente ragione. Poiché però nella giornata di oggi si è detto addirittura che non volessimo votare,

sui quali abbiamo discusso oggi relativamente al decreto legislativo n. 106. La prevede che almeno venga fatta salva la possibilità da parte del procuratore di comunicare al Consiglio superiore della magistratura eventuali variazioni nell'organizzazione dell'ufficio stesso. stesso. In questo modo diamo tempo ai procuratori capo di organizzare, ai sensi del decreto legislativo n. 106, che ricordo è in vigore, il loro ufficio e poi darne comunicazione al CSM. Vorrei però segnalare l'attenzione soprattutto dei colleghi della Casa delle Libertà su un punto che mi sta colpendo e mi fa meditare su come stanno andando i lavori dell'Assemblea.

sembrava di essere in guerra e tutto si svolgeva tra urla e insulti da parte dell'attuale maggioranza nei confronti del Ministro e nei confronti anche del Presidente del Consiglio. *(Applausi dai Gruppi*

con l'Aula e con i colleghi, ma accanto al senatore Strano, se non sbaglio, c'è una borsa e sotto di essa una scheda disattesa.

possa essere accordata o relativamente condivisa solo per una minima parte dell'articolo, chiedo che venga approvato il rinvio solo

per l'impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti da parte del procuratore della Repubblica. L'emendamento 1.404 limita la dilazione ed il rinvio temporale

è stata proposta esclusività nella sospensione dell'efficacia, riguarda l'attività di vigilanza del procuratore generale presso la Corte d'appello, ritenendo che anche in questo caso la limitazione della sospensione, solamente della parte così normata in applicazione della legge delega e del decreto legislativo, possa non essere lesiva dell'impianto complessivo del decreto legislativo proprio in applicazione della legge delega.

2006, n. 109. Sostanzialmente, le proposte formulate sono di spostare a date alternative, allo scopo di dare una possibilità di scelta all'Aula parlamentare,

alla sospensione dell'efficacia dell'articolo 28 del decreto n. 109, solamente nelle parti richiamate

Il testo dell'articolo 28, comma 1, capoverso Art 11, secondo ed ultimo periodo, tratta del magistrato decaduto dall'impiego e dell'applicazione

La sospensione della normativa verrebbe, a nostro giudizio, ad inficiare la richiesta di una magistratura preparata secondo determinati criteri. Con questo emendamento chiediamo di sospendere l'efficacia del comma 6 dell'articolo 6, in cui si dice che la mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura. Noi pensiamo che

invariate, pur con un criterio prudenziale. Se vogliamo mantenere un minimo di interlocuzione con il Consiglio superiore della magistratura, siamo disponibili a rinviare tale termine.

con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano determinate le indennità spettanti ai professori universitari componenti della commissione. Questo attiene al compenso. di tale comma, sia assolutamente possibile in un momento in cui tutti sono chiamati a intervenire per ridurre il bilancio.

Dichiaro chiusa la votazione. **Il Senato non approva.**

posti vacanti nella funzione della magistratura giudicante. A noi sembrava più che legittima l'attuale impostazione che non avrebbe necessitato di alcun

per la possibilità di operare una mutazione di funzione. È una norma che addirittura agevola addirittura agevola la scelta dei magistrati ed introduce il criterio dell'anzianità: chi si trovava in servizio e aveva più di tre anni e ha fatto questo tipo di scelta dovrà essere considerato con un occhio di riguardo. Noi proponiamo che questa norma rimanga in vigore o che comunque non venga sospesa oltre il 31 marzo 2007, anche perché è stato singolare vedere il Governo presentarsi in Aula con un provvedimento che chiede quantomeno che tutto slitti al prossimo marzo; e, probabilmente, nel pensatoio delle Commissioni si ritiene che il margine di garanzia debba essere ulteriormente dilatato, spostando tutto

con le motivazioni che abbiamo letto - e che non condividiamo, del resto - nel decreto che ci viene posto. Presidente, quello delle sedi disagiate è un tema che ci è particolarmente caro, tant'è che nel documento programmatico del nostro partito, proprio con riferimento alla situazione particolare che talune aree del Paese soffrivano per l'oggettivo disagio delle sedi giudiziarie, abbiamo scritto un'articolata relazione. Ora, francamente, immaginare, cioè, che si debba sospendere anche questa norma, che incide su un problema certamente sensibile e fortemente avvertito da tutti coloro che hanno veramente a cuore

è totale; ne prendo atto. Però, vede, la materia che stiamo discutendo, i temi che stiamo trattando impongono la massima attenzione ed impongono che resti traccia, nei verbali dei nostri lavori, della nostra determinazione su questo argomento. Non è possibile che chi viva il disagio di un tribunale di frontiera poi non debba avere un beneficio; che chi ha occupato postazioni difficili, chi è stato a contatto con aree particolarmente complesse della società non debba poi beneficiare di una condizione particolare. Perché questa corsia privilegiata deve essere inibita? Io me lo chiedo e lo chiedo all'Assemblea. Mi meraviglio che l'atteggiamento o le scelte della politica debbano incidere su un fatto che oggettivamente è di una chiarezza assoluta. Tutti quanti diciamo di avere a cuore le sorti della magistratura; tutti quanti diciamo, con argomenti diversi, di voler intervenire per rendere migliori le condizioni di questa categoria benemerita, alla quale tutti siamo grati per l'impegno che spiega quotidianamente per tutelarci e per garantire la legittimità. Ebbene, ora si costituisce una condizione particolare per premiare proprio coloro che sono gli ultimi, perché i più disagiati, coloro che hanno scelto di servire la collettività in condizioni obiettivamente compromesse, perché c'è difficoltà di viabilità o c'è difficoltà dal punto di vista degli ambienti con i quali si interloquisce. Ci sono sedi in cui nessuno vuole andare, signor Presidente; eppure quel grande servizio sociale che è la giurisdizione, l'esercizio della giurisdizione, il rispetto della giustizia, e l'applicazione dei principi fondamentali, lì viene realizzato grazie a questi personaggi benemeriti. Allora, per quale ragione non dobbiamo tutelarli? Mi interrogo perplesso, signor Presidente, di fronte all'atteggiamento del Governo e del relatore e li invito a riconsiderare l'opinione che hanno espresso su questo argomento.

questo segmento limitato, questi pochi ed eroici uomini della magistratura non debbono beneficiare dell'attenzione maggiore da parte del Parlamento repubblicano?

la copertura delle sedi disagiate rappresenta un momento particolarmente difficile dell'esercizio completo e concreto della giurisdizione, in particolare con riferimento ai posti di secondo grado. Infatti, le sedi disagiate di primo grado possono comunque periodicamente essere coperte con gli uditori giudiziari che, a volte anche *obtorto* *collo*, sono costretti ad accettarle; quindi comunque è assicurata una copertura periodica per questo tipo di sedi. Per sedi disagiate si intendono, tecnicamente, le sedi per le quali non è stata fatta domanda di trasferimento, secondo i bandi che ordinariamente vengono pubblicati pubblicati dal Consiglio superiore della magistratura, per un certo numero di occasioni. A volte sono sedi disagiate anche ridenti cittadine che non hanno nulla a che vedere con luoghi negativamente noti per una forte presenza di criminalità organizzata, ma per essere lontani dalle grandi vie di comunicazione e quindi dalla possibilità per il magistrato di avere poi anche una vita normale. Il problema però si pone in maniera particolarmente pesante per le sedi di secondo grado, per le quali è vero che è previsto anche un trasferimento d'ufficio, ma questo non viene mai azionato dal Consiglio superiore della magistratura, ovvero viene impugnato regolarmente davanti ai tribunali amministrativi e c'è una giurisprudenza costante di sospensione di questi provvedimenti che alla fine porta concretamente all'impossibilità di coprire le sedi disagiate, in particolare di secondo grado, perché in quelle di primo grado andranno gli uditori, più o meno *obtorto collo*, perché possano essere comunque coperte. Nel momento in cui comunque riusciamo ad avere dei magistrati che hanno richiesto certamente anche contando su quelli che possono essere i vantaggi della situazione di coprire un posto in una sede disagiata - perché anche questo tipo di vantaggi consente di far sì che anche in queste sedi possa essere amministrata la giustizia e che comunque vi possa essere un corrispettivo per i disagi che il magistrato incontra - sarebbe per lo meno incongruo prevedere una sospensione analoga a quelle delle altre norme dei decreti delegati dell'ordinamento giudiziario e cioè a luglio 2007, quando costoro hanno già messo in conto la possibilità di poter rientrare, dopo quel periodo che hanno deciso di trascorrere nella sede disagiata. S'impone certamente una differenziazione nelle date di sospensione, perché ci troviamo in una situazione particolare e specifica, se facciamo di tutta l'erba un fascio penalizzeremo questi magistrati che comunque sono andati a svolgere un ruolo con tutte le difficoltà possibili e immaginabili. è necessario graduare e modulare diversamente la sospensione e d'altra parte la data del 31 marzo 2007, tutto sommato, corrispondeva all'indicazione originaria di partenza delle sospensione delle norme sull'ordinamento: perché allora penalizzare questi magistrati? La mancata approvazione dell'emendamento 1.421 significherà voler penalizzare coloro che vanno in queste sedi disagiate, vorrà dire alla maggioranza e al Governo non interessa che si siano fatti carico di questa necessità di copertura, che li tratteranno esattamente come gli altri. Tutto ciò evidentemente non è pensabile, non è possibile. Bisogna operare una differenziazione in virtù di una distinzione complessiva delle situazioni, non possono essere penalizzati

fondi al Ministero della giustizia operato dal cosiddetto decreto Bersani. Prima si diceva che mancava la carta quando il centro-destra aveva non solo mantenuto, ma addirittura aumentato le risorse a disposizione del Ministero della giustizia; certo, per ragioni di logica

dev'essere affrontata con molto realismo. Non è sede disagiata quella in cui vi sono particolari condizioni di malessere della giustizia. Sede disagiata, secondo l'ordinamento giudiziario e l'applicazione dei magistrati, è quella determinata sede per la quale non si trovano magistrati che chiedono di andare ad occuparvi posti. Pertanto, le sedi Pertanto, le sedi disagiate costituiscono spesso un dato casuale. Molto spesso sono anche un dato terrificante che indica la mancanza di magistrati in posti centrali. Voglio fare soltanto un riferimento di carattere territoriale e storico, perché ci si possa rendere conto della gravità della situazione. Come ha ricordato il senatore Centaro, mentre i giovani magistrati che escono dal concorso, dopo l'uditorato (molto ridotto, soprattutto negli ultimi tempi), possono essere mandati in qualsiasi sede,

vi è una zona nel nostro Paese in cui alto è il tasso di impunità e altissima l'infiltrazione criminogena. Mi riferisco alla Locride. Se vi andate a leggere la storia del tribunale di Locri, vi renderete conto che è un tribunale cronicamente disagiato. Lì vengono mandati magistrati che, per farsi le ossa e costituirsi un titolo nel futuro, si vanno a sacrificare. È una situazione drammatica. Quando leggo che a Locri - per esempio, a proposito dell'omicidio Fortugno - vi è una cattiva risposta da parte dell'organizzazione giudiziaria, è bene che si sappia che vi sono giovani che si sono sacrificati per andare lì e che soltanto l'anno scorso su 24 omicidi ne sono rimasti non scoperti 22. È una zona in cui il disastro e la diseconomia che si raggiunge fra politica e perversione della pubblica amministrazione hanno fatto sì che a Locri vi sia il tribunale con il più alto numero di cause previdenziali in Italia: oltre 22.000. Non possiamo punire questi magistrati, che scelgono volontariamente di andare ad occupare una posizione di trincea,

Signor Presidente, onorevole Ministro, care colleghe e colleghi, oggi sono molto contento perché finalmente si vota. È un avvenimento mondano qui al Senato con le fiducie poste per strozzare i dibattiti. Ho ascoltato i colleghi che hanno affrontato questo tema.

nelle loro capacità di analizzare i problemi posti alla loro attenzione, qui e fuori di qui. Ammetto l'addebito, ma non faccio parte anche di questo tipo di soggetti.

se in quest'Aula c'è una dialettica e, finalmente, un tema come questo è portato all'attenzione di tutti, non per motivi politici, ma per una valutazione soggettiva e oggettiva di difficoltà di soggetti che hanno fatto una scelta in base alla trovano una condizione per cui una proroga più allungata potrebbe essere penalizzante, mi chiedo, onorevoli colleghi di parte avversa, per quale motivo dovremmo essere avversi su questo punto, se non per una questione di schieramento. *(Applausi dal Diciamo la verità, è inutile che ci arrivino dagli altissimi sogli inviti a discutere, a chiacchierare, a confrontarci e a stabilire, su certi punti almeno, una consonanza quando non c'è una differenza che militi per una coerente posizione politica che io rispetto e che, anzi, amo, perché il Parlamento è l'organizzazione del dissenso, non del consenso. Il consenso può arrivare se c'è un'intenzione comune di capire il problema e di non opporsi per principio. Allora, io che ho ascoltato i colleghi, non intendo aggiungere nulla a quello che hanno detto, con la diversa esperienza che hanno su vari campi, tanto nella vita professionale, quanto nella precedente attività che hanno svolto. Io che ascolto queste affermazioni e quindi mi sono convinto con le loro dichiarazioni, chiedo a voi, amici colleghi della maggioranza, che**,** almeno su questo punto, vi possa essere una valutazione che non sia manichea, di schieramento, che non ci obblighi a consumarci il dito per votare, ma ci costringa qualche volta a far funzionare il cervello e, auspicabilmente, la coscienza.

se in qualche modo ho proferito verbi o pensieri poco rispettosi nei confronti dell'Associazione nazionale magistrati o dei magistrati.

alcune frange, peraltro autorevoli (stiamo parlando del segretario dell'Associazione nazionale magistrati), interpretano la separazione dei poteri in questo nostro Paese

Ritengo che siamo tutti d'accordo, maggioranza e opposizione, se dico che, comunque, proseguiremo il nostro dibattito come abbiamo fatto fino ad ora, parlando liberamente, nel massimo rispetto di tutti, senza aver paura di nessuno.

credo che egli debba dire qualcosa di fronte ad un magistrato che interviene così pesantemente nei lavori dell'Aula.

mi sembra di tornare a quando alcuni di noi ci trovavamo in Commissione bicamerale

svolgere. Signor Presidente, le ingerenze dell'Associazione nazionale magistrati sull'attività legislativa del nostro Paese sono state, e purtroppo continuano ad essere, sotto gli occhi di tutti.

Non esageriamo, colleghi,

Dico loro che il principio della separazione dei poteri è principio sacro e inviolabile della Costituzione. Non è un principio che tutela le maggioranze e le opposizioni, ma la democrazia del nostro Paese.

di un voto liberamente espresso in piena autonomia, senza condizionamenti, senza infingimenti, senza dichiarazioni esterne che possano incidere sui processi di valutazione dei singoli parlamentari. Dimostriamo che noi singoli parlamentari, al di là delle appartenenze politiche, abbiamo una coscienza ed un cuore che batte secondo le nostre opinioni e che non ci lasciamo condizionare da certa magistratura che vuole invadere una competenza che non le appartiene.

Mi associo alla richiesta del collega Matteoli nei confronti del Ministro e del collega Schifani nei confronti di tutti i membri di questo Senato. Io credo che, di fronte a questa presa di posizione, sia indispensabile una presa di posizione netta del Presidente del Senato che ribadisca la sovranità del Parlamento quale espressione della sovranità del popolo e che difenda le nostre prerogative di Parlamento rispetto a questa invasione di campo, ancora una volta una travalicazione, un tentativo di costituirsi in partito da parte di quelli che dovrebbero essere servitori dello Stato. *(Applausi

Adesso sto parlando io. Testimonio il clima di assoluta serenità e tranquillità, tranne la prima fila che disturba - e devo testimoniarlo

però, senatore Castelli, non so quello che abbia detto, perché lei ha parlato e gli altri hanno replicato. Io quindi sono testimone qua, fuori dall'Aula francamente non lo so.

Senatore Buccico, ieri non l'ho censurata per l'espressione «fottere» che ho messo tra virgolette perché riferiva cose dette da altri, ma adesso basta! Dichiaro aperta la votazione. *(Segue la votazione).*

Presidente, quello che è accaduto era stato già prefigurato in uno degli ultimi interventi della seduta scorsa. Presidente, mi lasci introdurre l'emendamento; è soltanto una frase introduttiva per dire che... Il presidente Cossiga aveva lanciato un appello a quest'Aula dando una specie di linea di condotta: sempre, sempre, sempre contro l'Associazione nazionale magistrati. Questo era il monito di Cossiga; non contro la magistratura, contro l'Associazione nazionale magistrati,

L'Associazione nazionale magistrati ha perfettamente ragione, perché le norme di cui stiamo parlando sono veramente eversive, sovversive! si introduce il concetto - me lo consenta, Presidente - secondo il quale il Consiglio superiore della magistratura valuterà i magistrati in base alla loro laboriosità:

di questa misura tramite i decreti adottati dallo scorso Governo. Ma se facciamo un passo indietro, dobbiamo ricordare le grandi battaglie fatte proprie dalla sinistra per introdurre il concetto dell'operosità nella pubblica amministrazione, che è la meritocrazia. Come applichiamo la meritocrazia al settore della giustizia se non si può intervenire a fare valutazioni di merito? Questo emendamento è legato anche al concetto della funzionalità degli uffici o, meglio, della temporaneità della direzione degli uffici.

dell'entrata in vigore. Ma se continueremo ad accettare questo comportamento dell'Associazione nazionale magistrati, la prossima richiesta che perverrà sulla sua scrivania sarà lo stralcio di questo emendamento. Allora, Presidente, parleremo successivamente, quando si porterà